sta per concludersi l'anno europeo delle pari opportunità e siamo costretti a rilevare che l'Italia, il Governo italiano, non ha certamente brillato per iniziative e progressi nell'ardua marcia delle donne verso la compensazione del *deficit* di genere. Dico subito che questa mozione, che con le colleghe senatrici di maggioranza e di opposizione è stata presentata all'attenzione dell'Aula il 19 febbraio scorso e successivamente alla stampa, non fa eco a superate rivendicazioni sessiste, ma prende atto, viceversa, di una situazione assai grave che si sta verificando proprio per un eccesso di presenza femminile sui *mass media*, presenza quantitativamente, e non qualitativamente, apprezzabile, che di fatto compromette il difficile cammino della donna verso l'autorevolezza. I mezzi di comunicazione di massa, ma ci riferiamo in questo caso in particolare al servizio pubblico radiotelevisivo, pur essendo d'obbligo un onesto distinguo tra radio e televisione, ci stanno proponendo uno stereotipo di donna che non aiuta certo la crescita culturale delle giovani generazioni. Nonostante le donne abbiano raggiunto posizioni di livello in ambito professionale, sociale, artistico e culturale, il loro ruolo e la rappresentazione della loro immagine nei *mass media* rappresenta ancora, ma forse è più corretto dire sempre di più, vista la crescente degenerazione del sistema, un punto critico sul quale sono necessarie più profonde riflessioni in direzione di una radicale riqualificazione. Si tratta, in sostanza, di decostruire un modello e costruirne uno più rispondente alla realtà dell'impegno maschile e femminile di questi ultimi anni verso le pari opportunità. L'Italia vanta un sistema di norme assai garantiste a favore della donna che lavora, ma queste norme sono troppo spesso aggirate e disattese; analoghe garanzie legislative non si riscontrano in tema di partecipazione parlamentare ed alla vita pubblica, anche se questa legislatura deve imporsi di affrontare il tema nella riforma elettorale. Il punto più basso, comunque, la donna lo vive, quotidianamente e spesso inconsapevolmente, proprio nei luoghi e apparati di formazione dell'opinione pubblica e pratica culturale, non tanto in ordine alla visibilità, a mio parere attualmente sovradimensionata, ma segnatamente in ordine alla qualità dell'immagine fornita. Già nel 1985 la Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sulla condizione femminile, svoltasi a Nairobi, aveva inserito il rapporto tra donne e *media* nell'elenco delle 12 aree tematiche critiche su cui intervenire. Il recente Libro bianco su «Donne e *media* in Europa», promosso nel 2006 dal CENSIS insieme all'Unione Europea e alle fondazioni Adkins Chiti e Risorsa Donna, dopo aver proclamato l'Italia insieme alla Grecia il Paese meno interessato al tema delle pari opportunità, mette in evidenza come appaia dai *media* un'immagine assolutamente falsata della realtà femminile. Dall'analisi effettuata nell'arco di un'intera settimana per 24 ore al giorno dei programmi delle reti RAI, MEDIASET e La7 si ricava un modello proposto di ragazza giovane, bella e patinata, associata quasi sempre alla moda e allo spettacolo. Un'immagine di donna oca e discinta, perennemente e ossessivamente ammiccante, che diventa un *topos* della comunicazione, e perciò solo apparentemente innocuo e futile, ma in realtà molto pericoloso perché «strutturante» dal punto di vista dell'antropologia culturale. La specificità del modello italiano, rivela il rapporto CENSIS, è l'evidente scadimento dell'immagine femminile in televisione, nella cartellonistica stradale, nella pubblicità, sui quotidiani e sui periodici. La *fiction*, rivela il rapporto, è invece il genere televisivo che più e meglio di tanti altri tenta di intercettare il cambiamento sociale che ha interessato l'universo femminile. Ma ovviamente non basta. Proprio la ricerca «*Women and media in Europe*» propone soluzioni e linee operative, quali la formazione e la sensibilizzazione degli operatori, l'autoregolamentazione e l'ideazione di campagne di comunicazione. Tutto ciò, lo riaffermo con forza, è mancato in questo Anno europeo delle pari opportunità nell'azione del Governo italiano e in particolare del ministro Pollastrini. Eppure il servizio pubblico radiotelevisivo ha segnato in questi ultimi anni, tappe importanti verso la parità dei rapporti e la rappresentazione della differenza di genere. Vorrei qui ricordarne sinteticamente e brevemente alcune. Nel 1987 viene costituita la Commissione pari opportunità della RAI fino ad arrivare al significativo ampliamento a tutte le strutture aziendali e regionali nel 2004. Nel 1997 la Commissione di vigilanza RAI approva l'atto d'indirizzo «Donne e trasmissioni televisive», che porterà alla circolare della direzione generale della RAI del 18 settembre 1997 e al «Progetto donna» di RAI International, realizzato in RAI su *format* sperimentali di programmi radiofonici. Nel 2001 si costituisce un *think tank* nella rete *Gender Portrait*, formato da operatrici ed esperte della comunicazione esterne ed interne alla RAI. Si fa strada l'idea che non basti più un gruppo di programmi, ma una struttura che dia stabilità e visibilità all'informazione qualificata sulla donna: il circolo Guidotti, interno alla RAI, chiede la formazione della struttura «RAI Donna». Nel 2003, nell'ambito della discussione in Parlamento sul riassetto del sistema radiotelevisivo, il Governo accoglie una serie di ordini del giorno volti alla creazione di una specifica struttura che produca programmi trasversalmente trasmessi su tutte le reti, che evidenzino il contributo artistico, culturale, scientifico e politico che le donne hanno dato nel corso dei secoli. Nello spirito della modifica dell'articolo 51 della Costituzione, che ci impone leggi ed azioni positive per favorire le pari opportunità tra uomini e donne, la mozione che ci avviamo a votare invita la RAI alla creazione della struttura «RAI Donna», a creare una testata giornalistica, televisiva e radiofonica e uno spazio *web*, e a potenziare i progetti già esistenti per le pari opportunità.

che questo obiettivo sarà raggiunto in prospettiva per quello che attiene alla struttura, e in un prossimo futuro per quello che attiene alle testate giornalistiche. Del resto, esistono in Italia precedenti illustri per quello che riguarda il settore giornalistico della carta stampata: i due maggiori quotidiani, il «Corriere della Sera» e «la Repubblica», hanno prodotto già da qualche anno due allegati che hanno le medesime finalità: la presentazione di un'immagine femminile più qualificata e vera, non stereotipata e commerciale; l'acquisizione della normalità della compresenza storica in campo artistico, culturale, scientifico, politico e sociale nell'ambito della visione e della ricezione del pubblico; la promozione, così come previsto nel citato atto di indirizzo della Commissione di vigilanza RAI, all'interno del sistema radiotelevisivo pubblico, dell'acquisizione di poteri e responsabilità delle donne per integrare il punto di vista della differenza di genere nell'ambito delle politiche aziendali e della programmazione dei palinsesti. Era infatti proprio la Commissione di vigilanza RAI che, in questo atto scarsamente applicato, auspicava il ricorso da parte della RAI ad un organismo tecnico di garanzia per la valutazione della rispondenza dei programmi ai criteri. Voglio, infine, solo sfiorare il tema caldo, acceso dal recente dibattito sviluppatosi sull'ipotizzata o verificata corruzione del sistema, che vedrebbe le lavoratrici femminili del mondo radiotelevisivo oggetto di pressante*mobbing*. Un ulteriore motivo di riflessione sul tema delle garanzie per le donne e sulle pari opportunità. Tutte queste facce di un unico problema impongono al sistema radiotelevisivo pubblico un'assunzione di responsabilità che possa essere trainante rispetto ad ogni altro tipo di realtà, privilegiando sempre la qualità. Non esageriamo nel porci come obbiettivo finale l'istituzione di un codice etico dell'utilizzo della figura femminile in televisione, nella cartellonistica e nella pubblicità. È ormai assai lontano quel 1978 in cui il *Focus Group*, il primo gruppo di ascolto spontaneo interno alla RAI, composto da programmiste, analiste e ricercatrici, iniziò a visionare e analizzare i programmi per comprendere quale percezione si ricavasse all'esterno del femminile. Ancora oggi informazione, *fiction*, pubblicità, intrattenimento e *reality* tendono a riportare l'evidenza del punto di vista maschile con le sue conquiste e i suoi primati culturali. Ecco perché non dobbiamo dimenticare che il mezzo televisivo, considerato giustamente il più pervasivo tra i mezzi di comunicazione di massa, non riflette solo la realtà, ma può amplificarla, condizionarla e distorcerla. Questo *gap* storiografico sarà colmato solo quando non si comunicherà più solo attraverso il corpo della donna, ma sarà comunicato il suo sguardo, la sua visione, in una parola la sua anima.

il problema della rappresentazione della donna nei *media* non è un problema che si possa più trascurare. Esso assume tanto più rilievo quanto più le donne acquisiscono competenze e assumono ruoli importanti nella società e nelle professioni. Rispetto a una domanda di *empowerment* femminile, di riconoscimento del nuovo protagonismo nella società, nei *media* c'è una risposta che tende a rappresentarla pressoché esclusivamente secondo un'immagine stereotipata, legata a ruoli subordinati e, soprattutto per quanto riguarda la pubblicità, al richiamo ossessivo alla perfezione fisica che crea, tra l'altro, non pochi problemi psicologici nelle giovani donne. Ha richiamato su questo l'attenzione anche il Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione TV e minori, sottolineando come il modo in cui la TV rappresenta la donna ha un effetto enorme sia su come lei percepisce se stessa in rapporto agli uomini e al contesto sociale, sia sulla percezione che delle donne gli uomini e i minori. È del tutto evidente l'effetto di questi messaggi - ripetuti all'infinito - sui bambini e sugli adolescenti: per i ragazzi, considerare la donna essenzialmente come un corpo; per per i ragazzi, considerare la donna essenzialmente come un corpo; per le ragazze, aspirare soprattutto ad avere un bel corpo da usare come arma di seduzione e come biglietto d'ingresso nel mondo dello spettacolo. L'immagine della perfezione estetica diventa un modello per tante adolescenti che ad esso si ispirano fino ad arrivare ad ammalarsi di anoressia. Riteniamo che questo sia il momento per operare una svolta, per richiamare tutti i *media*, ma soprattutto le televisioni, a un maggiore rispetto della dignità delle donne, a una rappresentazione più fedele della nuova realtà in cui agiscono le donne. Tutte le statistiche ci dicono che le donne oggi sono più istruite degli uomini, più laureate, più impegnate nelle professioni, nell'imprenditoria, nella produzione culturale; aspirano a essere padrone della loro vita, protagoniste nei settori in cui operano, non più sottomesse e in ruoli subordinati. Soprattutto, non accettano più di essere rappresentate secondo un'immagine stereotipata di una figura che si trova a suo agio solo nel ruolo di chi è preoccupato prevalentemente della sua immagine estetica in funzione della seduzione erotica. Chiediamo che possano emergere l'intelligenza e la creatività delle donne, le loro capacità intellettuali e d'innovazione. Le donne vogliono essere, non solo apparire. È necessaria un'iniziativa più forte ed efficace per promuovere una diversa cultura della comunicazione sulla donna. Questo è oggi il problema: una nuova cultura della comunicazione sulla donna che sia di promozione, di rappresentazione di una figura complessa, che è mutata nel tempo, è diventata soggetto consapevole delle sue libertà e dei suoi diritti, prima di tutto il diritto, previsto dalla nostra Costituzione, a non essere discriminata. C'è una moderna libertà femminile che chiede di essere riconosciuta e rappresentata anche nei *media*. L'indagine del CENSIS, già richiamata dalla collega Allegrini, che è stata svolta nell'ambito del progetto «Donne e *media* in Europa», ha dimostrato chiaramente che la TV fornisce un'immagine distorta della donna oggi, dei suoi problemi (che sono tanti e diversi), delle sue aspirazioni, delle sue consapevolezze. Il tema al quale le donne vengono per lo più associate, nel 38 per cento dei casi, è quello della moda e dello spettacolo, collegato di nuovo a quello della bellezza; sui temi della cultura le donne intervengono solo nel 6 per cento dei casi; su questioni che attengono alle professioni nel 2 per cento dei casi, per la politica nel 4,8 per cento dei casi. Una presenza rilevante viene poi occupata da episodi di cronaca nera e di violenza, purtroppo sempre più numerosi. Quando vengono chiamate in quanto esperte, le donne sono per lo più invitate a parlare di natura e di astrologia; quindi poco o niente per le donne che studiano, che si affermano nelle professioni e nelle attività creative, che fanno ricerca, che amministrano, che si occupano delle istituzioni. dunque, dimostrano chiaramente che le donne nei programmi televisivi hanno scarsissima voce. Come si dice nel rapporto CENSIS, «si parla di lei, ma non le si dà la parola». Ciò è sicuramente dovuto anche alla scarsa presenza di donne nei luoghi decisionali delle aziende televisive, negli spazi di approfondimento e nei ruoli di conduzione delle trasmissioni, che sono ancora in grandissima parte nelle mani di uomini. Ma la ragione vera della rappresentazione distorta dell'immagine femminile nei *media* è frutto anche di una cultura che conserva ancora tratti patriarcali nella concezione del rapporto fra i due generi, che consente un uso consumistico del corpo e dell'immagine della donna, oscurando le nuove realtà e le nuove culture che le donne hanno costruito nel tempo. Questo 2007 è l'Anno europeo delle pari opportunità. Molte iniziative sono state prese anche per combattere le discriminazioni di genere, che sono ancora tante, troppe e riguardano il lavoro, i salari, la rappresentanza istituzionale e politica, il ruolo sociale. Se perciò noi chiediamo a questo Governo di dedicare più attenzione al problema delle donne nei *media* e sui *media*, è perché siamo convinte che, nonostante documenti importanti di istituzioni nazionali e internazionali come il Consiglio d'Europa, l'ONU - che da tempo hanno posto il problema, nel corso degli anni poco o niente sia stato fatto e - soprattutto - lo chiediamo a questo Governo, perché siamo convinte che un modello stereotipato non solo sia lesivo della dignità delle donne, ma nuoccia alla loro possibilità di affermazione sociale negli ambiti in cui aspirano a realizzare la loro personalità, nelle professioni e nelle carriere. È davvero auspicabile, dunque, che in questo Anno europeo delle pari opportunità il Parlamento, il Senato, dia un segno di volontà di svolta e che il Governo assuma tutte le iniziative utili, come ha cominciato a fare con altri temi, come la violenza sessuale. Chiediamo al Governo di assumere le iniziative necessarie affinché il sistema radiotelevisivo pubblico svolga un'opera di sensibilizzazione al rispetto della diversità di genere e della dignità delle donne, finalizzata ad una corretta rappresentazione della figura e del ruolo delle donne e alla rimozione di espressioni di discriminazione degli stereotipi lesivi della sua dignità; di promuovere campagne di informazione finalizzate alla diffusione e alla valorizzazione del lavoro e delle opere delle donne in campo artistico, culturale, scientifico e politico, e ad adottare campagne di sensibilizzazione nelle scuole, e in particolare nella scuola secondaria, per aiutare i giovani a rifiutare i messaggi discriminatori nei confronti delle donne ed evitare il perpetuarsi di stereotipi che danneggiano le donne e il ruolo femminile nella società; e ancora, chiediamo al Governo di promuovere l'acquisizione di poteri e responsabilità da parte delle donne in tutti i settori della vita produttiva e sociale, in particolare nell'ambito dei *media*, con azioni antidiscriminatorie mirate, per il reale accesso delle donne alle posizioni dirigenziali nel sistema radiotelevisivo pubblico al fine di favorire la presenza femminile nelle posizioni apicali delle testate giornalistiche televisive pubbliche, e più in generale del sistema radiotelevisivo pubblico, e di incidere sulle scelte editoriali e di palinsesto e quindi sull'immagine complessiva delle donne offerta dalla televisione pubblica. Noi, signor Presidente,

le mozioni nn. 61 e 136 presentano spunti rilevanti e suggeriscono linee di intervento che il Governo condivide e sulle quali fonda una componente importante della propria identità. Nello specifico, la recente stesura del nuovo contratto di servizio tra Stato e RAI ha dato una significativa prova della nostra determinazione in questo senso. Nell'articolo 2 del contratto, che ne stabilisce l'oggetto definendo la specifica missione del servizio pubblico, è inserita tra i compiti prioritari la valorizzazione del tema della condizione femminile e delle pari opportunità. Nell'articolo 4, che definisce l'offerta radiotelevisiva e in particolare alla lettera *c)* del primo comma, si prevede che le reti generaliste terrestri riservino un'ampia percentuale della programmazione a «trasmissioni finalizzate a comunicare e a valorizzare una più moderna rappresentazione delle donne, con particolare attenzione alla loro crescita sociale, ai loro diritti costituzionali e al loro ruolo nella società civile, nelle istituzioni e nel mondo del lavoro». Già questo segna una discontinuità importante, che è resa ancora più significativa dal fatto che queste disposizioni si accompagnano, nel contratto di servizio, alle previsioni di sedi e organismi investiti dell'«obiettivo di procedere (...) alla definizione delle più efficaci modalità operative di applicazione e di sviluppo delle attività e degli obblighi previsti nel (...) contratto, nonché di verificarne l'adempimento». Ciò determina una discontinuità che si dimostrerà ancor più influente sul piano concreto, giacché potrà almeno ridurre di molto le cause che hanno spesso indotto osservatori e largo pubblico a ritenere le prescrizioni del contratto di servizio, su questo come su altri temi, lodevoli quanto vuote petizioni di principio. Se poi il disegno di legge sulla riforma della RAI, presentato dai Ministeri delle comunicazioni e dell'economia e assegnato a questo Senato, dovesse tradursi in legge in tempi congrui, come auspichiamo, aumenterebbero ulteriormente i mezzi in grado di arricchire l'articolazione dei fini e degli strumenti per l'attuazione della missione autentica del servizio radiotelevisivo pubblico, e crescerebbe la loro efficacia. Le donne in carriera, nel settore della comunicazione in generale, raggiungono sempre più spesso i vertici della piramide. Oggi, circa il 77,8 per cento dei dirigenti dell'area comunicazione e il 55,6 per cento dei responsabili degli uffici stampa sono donne, nel 2002 erano, in entrambi i casi, solo il 38,9 per cento. Questi i dati che emergono dall'indagine «Donna e Comunicazione: valore e trasparenza» realizzata dal CENSIS per la fondazione «Marisa Bellisario». Si tratta di una vera e propria peculiarità di questo settore rispetto ad altri dove è ancora forte la predominanza di uomini. Dalla direzione generale (77,8

- nei ruoli di vertice, quali consigli di amministrazione, presidenti, amministratori delegati, direttori generali. Il *trend* della *leadership* femminile *tout court* lascia comunque ben sperare. In tutte le direzioni aziendali, infatti, la presenza femminile dal 2002 ad oggi ha guadagnato terreno. E se la scalata a settori come produzione o ricerca e sviluppo avanza lentamente, le donne hanno fatto grandi passi avanti nel *marketing*,

Nel servizio pubblico radiotelevisivo non possiamo dire che la situazione sia rosea, ma certamente è in atto un processo esplicito di affermazione femminile nei ruoli di vertice. Se si guarda all'organico RAI di oggi risulta immediatamente evidente una presenza femminile significativa, benché nei ruoli intermedi, sia giornalistici che amministrativi, il rapporto donne-uomini sia di uno a due, mentre nei ruoli dirigenziali il rapporto scenda ad uno a tre. Ma non possiamo dimenticare che nella storia non più brevissima della RAI ci sono state già due donne presidenti del consiglio di amministrazione (Moratti e Annunziata), due donne direttori di testata (Brancati e Annunziata) e attualmente una donna vicedirettore di RAI 1, una donna direttore della testata «RAI Parlamento» (Giuliana Del Bufalo), una donna direttore di «RAI Teche» (Barbara Scaramucci). Per ciò che attiene alle specifiche sollecitazioni che queste mozioni pongono, oltre ad esprimere la nostra piena condivisione dei loro obiettivi, tengo a sottolineare che l'impostazione che il Governo vuole dare a questo tema è quello di un'armoniosa integrazione di tali finalità nell'attività formativa e culturale del Paese, perlomeno per la parte sulla quale il Governo stesso ha voce in capitolo. Non condividiamo affatto l'idea che le donne, l'immagine e il ruolo femminili debbano essere oggetto sociale separato per la politica o addirittura obiettivi di una prescrizione di contenuto da parte di un'autorità superiore. Anche nel contratto di servizio emerge chiaramente la volontà del nostro Ministero di non assimilare in alcun modo ciò che concerne la condizione femminile e le pari opportunità alla tutela di minoranze, né a imporre una prefigurazione di ruoli calata dall'alto, tanto meno quando si tratti di ruoli ancillari e subordinati, per quanto li si possa poi rivestire di tratti leggiadri e amorevoli. Non pensiamo che la donna debba essere confinata in un'area protetta, ma separata: ogni azione contro la discriminazione o rappresentazioni fuorviate fuorviate e riduttive parte per noi dal principio che la diversità di genere e la presenza femminile rappresentino un fattore costitutivo della società italiana, che sta al cuore del suo corpo principale e non ha alcun motivo di essere relegata a una dignità periferica benché custodita. Da questo punto di vista ci pare di cogliere negli impegni indicati dal dispositivo della mozione che ha come prima firmataria la senatrice Allegrini una caratterizzazione un po' da «orto chiuso» (che mi sembra in ogni caso superata) o comunque da ambito separato, in contrasto con la filosofia che ho sopra esposto e con i passi concreti che essa ha finora ispirato: passi che difficilmente si potrebbero definire timidi o inconcludenti rispetto a quelli compiuti in analoga sede nel corso della legislatura precedente. Naturalmente molto resta da fare, a cominciare dalla attuazione dalla verifica puntuale di quanto già previsto. Oltre a tali precisazioni, è necessario qui puntualizzare - anche in relazione al terzo impegno indicato nel dispositivo della mozione di cui Franco - che il nostro parere favorevole rispetto agli impegni previsti dalle mozioni è tuttavia sottoposto a un'importante condizione, ovvero il limite posto dalle norme alla sfera di intervento autoritativo del Governo, in particolar modo per quel che riguarda le scelte gestionali dell'azienda RAI e l'autonomia della medesima nell'elaborazione delle forme più opportune per dare attuazione editoriale agli obiettivi posti dal contratto di servizio. La richiesta circa la necessità di favorire la effettiva acquisizione di potere e responsabilità attraverso l'accesso alle posizioni dirigenziali nell'ambito della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo non può prescindere dalla normativa vigente in materia, in particolare dall'articolo 3 della legge n. 206 del 1993 (tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 20 della legge n. 112 del 2004) che, come è noto, pone in capo al direttore generale della RAI la competenza riguardante sia la nomina dei dirigenti di primo e di secondo livello, che è proposta al consiglio di amministrazione, sia l'assunzione, la nomina, la promozione e la collocazione di dirigenti, nonché, su proposta dei direttori di testata e nel rispetto del contratto di lavoro giornalistico, degli altri giornalisti. L'attività di sensibilizzazione e promozione delle pari opportunità spetta alla comunicazione delle istituzioni. Compete quindi al Governo la promozione di ogni tematica di rilevanza sociale, a cominciare dalla questione femminile. valorizzare le differenze, promuovere la conciliazione, delineare percorsi professionali che tengano conto anche dei tempi delle donne. Poche le iniziative già portate avanti negli ultimi anni: il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nel 2005, ha diffuso un opuscolo informativo sulla possibilità di usufruire di permessi speciali nel caso di tumore al seno. Il Ministero delle pari opportunità si è occupato, oltre ad altre questioni, di quote rosa e violenza sulle donne. Ma è mancato fino ad oggi un impegno esplicito di sensibilizzazione contro le discriminazioni sul lavoro, a favore di un pieno riconoscimento dei diritti delle lavoratrici, in particolare nel momento della maternità. Allo stesso modo si ritiene necessario favorire l'affermazione, attraverso finanziamenti specifici, di una comunicazione di genere a livello regionale e locale, traendo spunto da alcune esperienze già avviate con successo, per esempio in Piemonte. Impegni importanti che il Governo vuole assumere e per il quale sarà necessario prevedere adeguati stanziamenti di bilancio a favore del Dipartimento per l'informazione e l'editoria che dovrà curare la realizzazione delle campagne. In questo ambito sarà rilevante anche l'impegno dell'azienda di servizio pubblico radiotelevisivo che ha la possibilità di entrare con il messaggio all'interno delle famiglie italiane. Sarebbe altresì auspicabile e possibile l'istituzione di un osservatorio delle donne nella comunicazione e nei *media*. Un osservatorio capace di monitorare la presenza, sia in termini quantitativi che qualitativi, delle donne che operano nel campo dell'informazione, dell'ICT, del mondo dell'audiovisivo e della pubblicità rispetto al quadro complessivo delle professioni. Secondo l'indagine del *World Economic Forum* che ha creato il *Gender Gap Index*, l'Italia risulta agli ultimi posti della graduatoria: quarantacinquesima su 58 Paesi rilevati, con l'aggravante di essere anche il fanalino di coda dei Paesi europei. L'osservatorio dovrebbe avere anche l'obiettivo di misurare la presenza in televisione delle donne in veste di esperte, studiose o protagoniste di *fiction*, rispetto alle donne attualmente protagoniste dell'*infotainment* (modelle, donne di spettacolo, giovani spesso belle e poco vestite), uno strumento per superare categorie e stereotipi inadeguati.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Sottosegretario, il Gruppo per le Autonomie voterà a favore di entrambe le mozioni. Mi si consenta di dire, alla luce anche delle impegnative conclusioni del Sottosegretario, che forse l'obiettivo è stato centrato.

Parlamento l'enorme problema non tanto e non solo dell'*empowerment* femminile in tutti i settori della vita associata, lavorativa, legislativa, della presenza nelle istituzioni di cui ben conosciamo le difficoltà, ma anche dell'immaginario, del simbolico, dei modelli e del messaggio potentissimo che influenza la cultura di massa. Immagine, percezione, modelli della donna sono il tratto di una civiltà e i *media*, particolarmente quelli radiotelevisivi e televisivi, sono il veicolo fondamentale, nei tempi contemporanei, di questo simbolico, di questa percezione e quindi, in ultima analisi, di questo condizionamento sui tratti della civiltà. Il problema non è la presenza femminile, ma il simbolico femminile, il modello di cultura di massa, come giustamente dicevano le senatrici presentatrici

di ciò che il Governo solleciterà, e ha attribuito una specifica funzione di autonomia e di responsabilità, come è giusto, alla RAI, ai suoi dirigenti e al suo direttore generale.

affinché non ci si rassegni più allo stato delle cose esistenti. La primissima interrogazione che presentai in Senato un anno fa riguardava la questione delle *soubrette*, delle vallette, dei dirigenti RAI impegnati in

un *curriculum* (la Regione Campania si era anche impegnata a pensare a qualcosa di simile), un albo, la possibilità di essere riconosciute, un *iter* professionale; chiedevo perché, nel mondo così importante dell'intrattenimento televisivo italiano,

il genere dell'informazione propriamente detta, dove qualche passo in avanti si è fatto, sia per il ruolo delle giornaliste, sia per i temi che l'informazione generalmente tratta, anche se qualche *deficit* nell'informazione sportiva, dove spesso il ruolo delle donne,

facciamo in modo che, per ciò che può, l'azienda pubblica dia il suo contributo a cambiare il Paese, a far entrare la vita delle donne - per quella che è davvero - nelle sue reti, ad avere l'ambizione di un'influenza culturale sulle nuove generazioni. Il tema che oggi il Senato ha tentato di affrontare non è il solito discorso sul ruolo delle donne:

Signor Presidente, signor Sottosegretario, colleghi, noi Comunisti Italiani e Verdi voteremo a favore delle due mozioni che hanno come prime firmatarie la senatrice Franco e la senatrice Allegrini, perché cogliamo come drammaticamente vera la constatazione in esse contenute, per cui la donna o è bella, maliziosa, vincente e spregiudicata o è vittima. Una lettura, questa, trasmessa in troppe occasioni dai *media*, inaccettabile per il suo carattere di vera e propria distorsione. Il nostro dibattito di oggi esemplifica come il mondo della comunicazione non sia neutro, ma contiene e aggrava i limiti e le contraddizioni della realtà, prima fra tutte la contraddizione di genere. Il tema dell'immagine delle donne nella comunicazione rende evidente un dato spesso sottaciuto, cioè quanto costa, in termini sociali, l'impari peso dei due generi. Il punto non è solo il diritto soggettivo delle singole donne, non è solo poter aspirare alla carriera che i propri meriti dovrebbero garantire; il punto è che l'informazione, lo spettacolo, la comunicazione, se fatti dai soli uomini, sono più poveri. L'inadeguata presenza delle donne nasconde esperienze, pratiche e condizioni di vita che solo loro possono raccontare in modo convincente. Si pensi all'enorme e delicato tema della procreazione oppure a come uomini e donne possono diversamente raccontare i propri tempi di vita. Una società che rifiuta le donne come soggetto del racconto collettivo della comunità non fa un torto solo alle donne, ma anche a se stessa. La distorta La distorta immagine femminile che ci rimandano molti palinsesti televisivi è il frutto dell'assenza delle donne, e della loro consapevolezza, dai circuiti delle decisioni. E l'effetto di questa assenza abbassa il livello della comunicazione italiana, che non è solo un mercato, ma una fonte educativa e uno dei principali legami sociali del Paese. Potremmo dire che questa assenza diseduca e immiserisce. Entrambe le mozioni che sono alla base della nostra discussione, con dati e citazioni, confermano il dato empirico: l'immagine femminile che i media e la televisione in particolare trasmettono è unidimensionale, ristretta, appiattita, come se le donne fossero solo quei corpi giovani e belli che si mostrano alle telecamere. Il punto non è negare in modo censorio che esista questo aspetto della realtà e una aspettativa distorta del pubblico, ma rifiutare che quella sia l'unica dimensione femminile possibile. Il tema che abbiamo di fronte non si risolve allora con un separatismo femminile, con la «televisione delle donne», come per esempio può auspicare qualcuno, ma con una rinnovata idea di pluralismo. Troppo spesso (e questo è un limite diffuso) si fa riferimento al pluralismo televisivo, come se il pluralismo si riferisse e si esaurisse in una sola dimensione, cioè quella della politica e delle appartenenze. E invece la difficoltà sta nell'unidimensionalità dei *format* televisivi e pubblicitari. Un mondo che parla di se stesso, che dimentica la realtà, che perde di vista le grandi questioni che appassionano e preoccupano gli italiani: lavoro, ambiente, famiglia, etica pubblica. Serve allora uno slancio di pluralismo che sia anzitutto culturale e tematico. Se questo è lo stato della comunicazione, il ruolo delle donne dentro la macchina organizzativa dei *media* è la conseguenza. I sette direttori dei telegiornali delle prime sette reti televisive nazionali sono tutti uomini, e questo nonostante che dentro le strutture che producono comunicazione e informazione di donne ve ne siano tante e capaci. Ci sono nella tv, come nella scuola, negli ospedali e negli altri settori della società. È una situazione nota e diffusa: le donne fanno e sono meritevoli molto più di quanto sia loro riconosciuto. Ad una questione generale si deve rispondere allora con politiche generali rafforzando il *welfare*, aumentando le opportunità di lavoro per le donne e promuovendo la responsabilità di un sistema produttivo ancora troppo miope, come si è positivamente iniziato a fare con il bollino rosa per le imprese o le politiche per gli asili nido e le classi primavera. Ma c'è uno specifico nella questione della comunicazione ed è uno specifico che richiede più iniziativa. Se la valorizzazione della differenza produce pluralismo allora bisogna essere più coraggiosi ed è un coraggio che passa anche da qui, dal Parlamento, dal potere legislativo. In questi giorni, è in discussione la norma che riforma la *governance* della RAI e modifica i criteri di nomina del consiglio di amministrazione RAI: oggi nel consiglio di amministrazione c'è una sola donna su nove esponenti. Deve per forza continuare ad essere così? Da tempo discutiamo di produrre delle quote di salvaguardia della presenza femminile nella rappresentanza del popolo. Perché questo principio, per esempio, non potrebbe essere sostenibile anche per quel che riguarda la guida collegiale della più grande azienda culturale del Paese? Servono quindi una maggiore consapevolezza e una maggiore iniziativa del Governo e del Parlamento. Noi oggi sosterremo le mozioni in discussione, assumendo questo impegno di responsabilità anche per l'azione, domani, di legislatori.

Nel nostro Paese le donne sono più numerose degli uomini. Le giovani laureate e diplomate sono più numerose dei loro coetanei e si laureano e si diplomano con voti migliori; nei concorsi pubblici raggiungono qualificazioni e risultati migliori al punto da dover introdurre, in certi concorsi, addirittura le quote per gli uomini. Purtroppo, a percorsi di qualità e a studi di specializzazione non corrisponde un adeguato inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni. Ad oggi, nel nostro Paese il tasso di occupazione delle donne è del 45 per cento, dunque notevolmente inferiore rispetto a quello degli uomini, che è pari è molto lontano dall'obiettivo di Lisbona (ricordo che nel 2010 l'Italia dovrà misurarsi con i livelli europei). Attualmente, siamo il penultimo Paese europeo per tasso di occupazione femminile. Sono dati un po' vergognosi.

Il precariato è un grosso limite della nostra società perché oltre a non permettere ai soggetti (in questo caso alle donne) di costruire un progetto di vita - le tante scelte di maternità tardive che spesso non raggiungono un esito felice ci rimandano esattamente a questo un alto livello qualitativo del lavoro svolto, a causa delle esperienze interrotte e scarsamente capitalizzate, e costituisce una disarticolazione di quei rapporti sociali fondamentali per una coesione della società. Il precariato in RAI è un dato antichissimo. Possiamo dire che la RAI è stata *ante litteram* un bacino di lavoro precario, dunque di vecchia tradizione: ricordo i contratti di sei o di nove mesi

una rappresentazione delle donne voluta secondo modelli femminili antichi o falsamente moderni - che poi è la stessa cosa - e comunque stereotipati: la madre casalinga, la ragazzetta falsamente spregiudicata, la valletta, le "veline", le "letterine" - ne hanno parlato altre colleghe molto meglio di me - che enfatizzano l'antico ruolo della donna oggetto sessuale. Intendiamoci: la bellezza fisica, anche se non deve essere l'unico parametro e metro di valutazione, è cosa positiva, piace a tutti, tanto nelle donne quanto negli uomini e su questo non vi è alcun dubbio. Casomai, sarebbe da chiedersi perché sia rappresentata con un unico modello omologato e falsamente emancipatorio. Il punto è che questi prototipi e modelli sono connotati da caratteristiche che spingono - lo ha detto benissimo la collega Franco prima - soprattutto le adolescenti, ma anche le preadolescenti a comportamenti *borderline*. L'aumento dell'anoressia nelle adolescenti produce, ad esempio, la sospensione delle mestruazioni. È un tema importante, ne va delle loro future scelte di maternità.

di un rapporto malato con il proprio corpo, enfatizzato da modelli di *media* e televisivi. Riproporre ossessivamente questa immagine per un servizio pubblico, che tiene alla formazione ed al livello culturale,

Stiamo affrontando, tramite lo strumento delle mozioni parlamentari, un argomento molto complesso, cioè il rapporto tra donne e mezzi di comunicazione di massa, in particolare la televisione; quel mezzo che, per la sua forza comunicativa, la sua pervasività emotiva e la sua influenza sui processi cognitivi, contribuisce a costruire la percezione collettiva del mondo. La prima osservazione rilevante e condivisa da entrambe le mozioni, che scaturiscono dalle stesse fonti di ricerca e fanno riferimento, in particolare, all'indagine del CENSIS 2006, è che la vita reale delle donne non viene rappresentata nello spazio mediatico. Quella che classicamente viene definita la condizione delle donne è sistematicamente rimossa, travisata o confinata in programmi ed eventi straordinari. Nello spazio televisivo prevale l'immagine della donna oggetto e della "velina" che, magari, fa da contorno e spalla al conduttore maschile. Nei programmi televisivi di intrattenimento, persino nelle *fiction*, scompaiono le donne anziane, le donne povere, le operaie, le casalinghe, le malate, le disabili, le disoccupate, le casalinghe che fanno fatica a quadrare il bilancio e perfino la tanto esaltata, nella cultura corrente, figura della madre, è marginale perché impossibile da rappresentare nella sua fatica fatica quotidiana reale, quando deve conciliare scelte di vita personali con l'esigenza di una società sempre più mercificata e segnata dalla guerra e dalle esigenze del profitto. Oppure la donna è rappresentata come soggetto debole da tutelare, travolta dalla violenza familiare e da tragiche relazioni d'amore. Nelle immagini pubblicitarie (come quelle che mettevano in scena, mi sembra fino al mese di giugno, allusivamente una violenza collettiva di giovani uomini contro una bellissima e indifferente signora), il corpo femminile è muto ed è solamente oggetto dello sguardo altrui. Si perpetuano, quindi, stereotipi di genere che non corrispondono più alla vita reale che scorre nella nostra società, in cui le donne non sono più solo vittime, ma soggetti, autrici del proprio destino, lavoratrici, intellettuali artiste, ricercatrici, professioniste impegnate nella solidarietà internazionale. Insomma, sono donne che operano in tutti i campi. Nello spazio mediatico, quindi, non si rappresenta la forza, la ricchezza e la qualità delle donne vive.

è che in nessuna delle due mozioni si riconosce il debito culturale che dobbiamo al movimento delle donne. Tutte e due le mozioni sono percorse

ricollegarsi fosse un dato negativo, come se l'eco di questo grande movimento, che ancora vive nelle piazze di tutti i Paesi del mondo e anche nei testi perché è un movimento che produce anche

Ma allora, a mio parere, che cosa può determinare quel cambiamento che tutte le mozioni richiedono in modo in modo netto? La rappresentazione stereotipata non si modificherà se chi fa comunicazione di massa è un soggetto prevalentemente maschile o anche una donna fautrice della neutralità del linguaggio. Come afferma la giornalista RAI Marina Pivetta, dire "ingegnera" in televisione vale più di interi convegni sulla rappresentanza femminile. Bisogna lavorare, insomma, sulla soggettività. Bisogna relazionarsi con le modalità con le quali in Italia si è configurato il rapporto tra donne che lavorano in questo settore, in particolare le giornaliste, e l'onda lunga dei movimenti di donne nel mondo. Il giornalismo italiano ha subito un processo intenso di femminilizzazione. Le donne sono presenti ovunque, non solo nella moda, nello spettacolo e, come giornaliste, nella cronaca, ma anche nella politica e nella cultura. Le donne sono state anche *reporter* di guerra. Le abbiamo viste in varie collocazioni illustrare gli orrori della guerra irachena sotto le bombe di Baghdad. Hanno prodotto coraggiose denunce e interessanti servizi, che spesso hanno avuto come tema il punto di vista emerso da Pechino, quando i vari movimenti femministi nel mondo si sono riconosciuti e dichiarati come soggetti centrali che ricostruiscono le condizioni per fermare la guerra, perché la politica prevalga sulle armi. C'è dunque nei *media* una presenza femminile emergente, ma non sufficiente potere. L'emancipazione di tante non cambia l'ordine del discorso corrente, non spezza lo stereotipo, non costituisce libertà per altre donne. Analizziamo, per esempio, le donne nella filiera produttiva della comunicazione, a partire dalle giornaliste. Anch'io ho dati differenti da quelli che il Sottosegretario qui enunciava. Da un lato, vi è il grande aumento quantitativo del numero delle giornaliste: dagli anni Settanta ad oggi, si passa dal 10 al 30 per cento di giornaliste

della conduzione giornalistica e quindi non riescono a determinare una modifica profonda dell'immagine e del prodotto, che è ancora connotato da quella struttura patriarcale della società

non c'è moltissimo da aggiungere a questo dibattito. Le senatrici che sono intervenute in dichiarazione di voto hanno toccato, ognuna di loro, campi diversi di applicazione del tema che stiamo trattando stamattina grazie alla presentazione di queste due mozioni. La mozione della senatrice Allegrini e quella della senatrice Franco ci aiutano ad affrontare, sia pure con tanto ritardo, un tema che è diventato quasi emergenziale per la nostra cultura,

tutto il dispiegarsi del mondo della comunicazione e dell'intrattenimento, così come oggi si dice, che è parte integrante, ahimé il più delle volte prevalente, della cultura e della comunicazione che trasmette cultura nel nostro Paese. Alla senatrice Pellegatta, però, vorrei far notare come i direttori delle reti che lei ha citato, che sono tutti inesorabilmente uomini,

Le dirigenti, onorevole Sottosegretario, sono ahimé molto poche, così come molto poche sono le donne in altri ambiti dalla vita anche pubblica del nostro Paese. Senza guardare alle istituzioni, dove penso che siamo decisamente più arretrati del Botswana, anche nel nostro apparato dello Stato le donne dirigenti contano come mosche bianche, nonostante l'ingresso massiccio di donne nell'apparato pubblico avvenuto negli ultimi anni per due fondamentali motivi:

anche se io (la senatrice Pisa ha fornito numeri eloquenti ed interessanti al riguardo) non vorrei cadere nella trappola di confondere quanto di buono ha realizzato, dal punto di vista quantitativo, l'introduzione della flessibilità nel mercato del lavoro

che non mi piace definire semplicemente e banalmente *tout court* precari, sono percorsi occupazionali che hanno consentito a tante donne di entrare, anche se in forma minima, flessibile

La senatrice Brisca Menapace, che conosce i percorsi delle donne e la vita delle donne italiane da tanti e tanti anni, sa bene che noi prima di quella data, in quel mercato, se non in quello pubblico attraverso i concorsi, non entravamo e non ci inserivamo nelle aziende, nelle imprese e nel tessuto economico in virtù di qualche errore da noi stessi commesso negli anni passati. La grande tutela della maternità, ad esempio,

secondo me, meglio di tanti uomini (come abbiamo visto negli ultimi anni e forse anche in quelli passati) possono gestire quel gigantesco sistema che è la RAI. Non intendo approfittare della bontà e della grande qualità di questo dibattito per scadere nella definizione di una RAI "baraccona", dove quella precarietà, che la senatrice Pisa ha raccontato molto bene prima, è anche il frutto di scelte

e l'individuazione di un percorso dove molte cose possono essere fatte. Non so se esista quel corretto rapporto di autonomia tra Governo e RAI. Faccio atto di fede insieme alla senatrice Negri e dalla RAI, dal servizio pubblico che noi tutti sosteniamo e dal quale ci attendiamo almeno il ritorno di un servizio adeguato ai soldi che versiamo quando paghiamo il canone - e lo paghiamo in tanti - mi attendo semplicemente una vigilanza sui temi e sugli *input* culturali che ormai al suo interno rappresentano il pane quotidiano. La qualità delle trasmissioni RAI, nella sua prevalenza, è assai bassa

linea culturale: quella dell'intrattenimento fatto passare sul corpo e sulla pelle delle donne. Ciò ha determinato la scarsa qualità della RAI di questi ultimi anni

si tratta di scelte che rincorrevano logiche commerciali - se voglio trovare una giustificazione, ma non la trovo nemmeno in questo modo - in virtù dell'accaparramento della pubblicità. Non trovo altra spiegazione nel proporci continuamente programmi di qualità scadentissima che, come ho detto prima e non voglio ripetermi, pongono al centro di questa scarsa qualità l'utilizzo del corpo femminile per l'*audience* o per la raccolta pubblicitaria. Quindi, signor Presidente, penso che il nostro dibattito e la presentazione di queste mozioni (che sono due atti formali e impegnativi mi auguro per questo Governo, ma anche per tutti noi)

di quella cultura femminile che, invece, abbiamo perso. Non vedo le donne casalinghe in televisione, ma solo signorine che offrono di noi un'immagine talmente deleteria da costituire oramai una piccola emergenza culturale in questo Paese. Infatti, come ha spiegato bene la senatrice Capelli, ciò ha indotto una serie di conseguenze che pagheremo tra qualche anno e che stiamo già pagando dal punto di vista culturale: le nostre adolescenti e le preadolescenti, che venivano citate prima nel

filosofe nel nostro Paese che ci hanno aiutato a connetterci con un mondo di emancipazione femminile, spesso proveniente dagli Stati Uniti, da Oltreoceano e da altre parti del mondo (il caso di Camille Paglia credo che sia uno dei più sintomatici e paradigmatici). Tutto questo è motivo per me di soddisfazione. Non è affatto motivo di soddisfazione, invece, dover notare che queste due mozioni forse andavano discusse la prossima settimana, signor Presidente, quando probabilmente in quest'Aula affronteremo il tema della RAI nella sua globalità. Allora, forse, avremmo avuto maggior attenzione da quei colleghi uomini che, se oggi non sono in massa come in altre occasioni, è forse perché quel linguaggio non lo sappiamo condividere con l'altro genere. Pertanto, la prossima soddisfazione che mi auguro di vivere è che il linguaggio delle donne e dell'UDI, oltre ad appartenere alle tante donne che in questo Paese non sono rappresentate

di poter condividere con tutta la rappresentanza del nostro popolo l'emergenza della volgarità che passa attraverso il messaggio della televisione ed in particolare, per quanto a noi compete, della televisione pubblica. Contro questa volgarità dobbiamo combattere e oggi queste due mozioni ci aiutano a ripartire con il piede giusto.

Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, colleghe e colleghi, è l'amore per la libertà, il bene più grande per il quale nella vita si possono affrontare i più grandi sacrifici, e il rispetto per la dignità di una donna straordinaria che si è identificata con il suo popolo che hanno mosso me e ad altri 74 senatori di diversi Gruppi politici di maggioranza e di opposizione a portare all'attenzione del Senato della Repubblica, con una mozione presentata nei mesi scorsi e oggi aggiornata, la condizione di una delle donne più coraggiose del nostro tempo, Aung San Suu Kyi, premio Nobel per la pace nel 1991, da anni agli arresti domiciliari, e quella del suo popolo, il popolo della Birmania, a cui è stato impedito di vivere nella democrazia dopo il trionfo della Lega nazionale per la democrazia nelle elezioni del 1990 con l'82 per cento un popolo che c'è caro per la sua storia, la sua cultura, la sua sofferenza a causa della violazione dei diritti umani a cui è sottoposto dalla giunta militare al potere da più di 45 anni. Siamo certi che la nostra iniziativa corrisponda al comune sentire democratico dell'Italia, nella consapevolezza che il destino dell'umanità è uno solo e che la pace e il progresso dei popoli, di ogni popolo sono un bene per tutti. Questo è lo spirito e la lettera della nostra Costituzione che, all'articolo 11, ripudiando la guerra, promuove e favorisce le organizzazioni internazionali che assicurino la pace e la giustizia. Dal secondo conflitto mondiale in poi la pace e il diritto, i diritti umani fondamentali sanciti dalle Carte internazionali, sono la base della convivenza umana ma oggi nel mondo globale lo sono ancora di più. Non solo l'economia e i commerci ma i diritti universali, la libertà, l'autodeterminazione e la sovranità dei popoli rendono fecondi i rapporti internazionali, sviluppano l'interdipendenza tra i popoli e gli Stati, costruiscono i nuovi scenari geopolitici del mondo. Questa è la ragione fondamentale che ci spinge oggi a discutere qui, esprimendo la volontà del nostro Paese nel mondo di cui siamo parte, affinché i diritti umani fondamentali siano affermati ovunque e in particolare nei luoghi in cui sono più violati come la Birmania, di cui Aung San Suu Kyi è simbolo e speranza. Figlia dell'eroe nazionale Aung San, considerato il padre della Nazione, ucciso nel 1947 a 32 anni agli albori dell'indipendenza della Birmania, alla quale aveva dedicato la vita, Aung San Suu Kyi è da anni alla guida del movimento per la democrazia nel suo Paese, sacrificando a questo scopo gli affetti familiari più cari così da identificarsi con la storia del suo popolo e il suo anelito alla democrazia. Aung San Suu Kyi ha conosciuto e apprezzato la filosofia gandhiana della non violenza fin da bambina, in India, dove ha vissuto al seguito di sua madre ambasciatrice. Ha avuto una formazione cosmopolita: ha studiato ad Oxford, ha lavorato all'ONU, ha sposato un inglese ed ha avuto due figli dai quali è stata costretta a separarsi quando, tornata nel 1988 in Birmania per assistere la madre, si è trovata coinvolta nella lotta contro il regime militare e, in piena repressione, ha detto no all'offerta di andare in esilio preferendo restare nel Paese, detenuta nella sua casa senza possibilità di alcun contatto con l'esterno. In diverse occasioni in questi anni, e negli ultimi mesi in particolare, la stampa nazionale e internazionale e l'opinione pubblica mondiale hanno parlato di lei. Il 19 giugno scorso, in occasione del suo sessantaduesimo compleanno, nella città di Roma in Campidoglio e in altre parti del mondo si è manifestato l'auspicio della sua liberazione. Ma è l'intera situazione della Birmania ad essere all'attenzione del mondo ed anche alla nostra. La dichiarazione finale della IV Conferenza sulla Birmania delle Confederazioni internazionali dei Sindacati, svoltasi a Katmandu in Nepal, il 3 e 4 aprile scorsi, scorsi, con la partecipazione di *leader* e rappresentanti del movimento democratico birmano in esilio, dà conto dei rapporti dettagliati sullo stato della repressione del Paese, con particolare riferimento ai diritti sindacali e del lavoro,

della priorità assoluta nel bilancio nazionale alle spese militari, oltre che della mancanza di sostegno alle necessità elementari del popolo in materia di sanità e di istruzione. Noi sappiamo bene che la militarizzazione del Paese ha reso la Birmania un Paese poverissimo, senza ospedali, né scuole, né trasporti, senza protezione sociale, senza libera informazione, senza democrazia, senza libertà: un Paese carcere. La stampa italiana ci ha informato del fatto recentemente, la chiusura alle informazioni della Giunta ha impedito perfino, nelle settimane scorse, di portare aiuti nelle zone colpite dalle inondazioni. Sono giunte notizie, in questi giorni, di ulteriori arresti per le manifestazioni contro gli aumenti del gas e del diesel, e di condanne per sedizione di sei sindacalisti a 20 e 28 anni di carcere, con un processo a porte chiuse, per avere organizzato un seminario sui diritti dei lavoratori il primo maggio all'*American* *Center* dell'Ambasciata americana. Ma la solidarietà internazionale è forte. Proprio la settimana scorsa, il 7 settembre, è stato assegnato a Palermo il Premio internazionale «Padre Pino Puglisi» 2007 al sindacalista birmano Zaw Tun, che lo ha ritirato in nome del sindacato birmano FTUB. Era presente, tra gli altri, il Vice presidente di quest'Assemblea, senatore Gavino Angius. Inoltre, gli organismi unitari di CGIL, CISL e UIL del 12 settembre scorso hanno approvato un ordine del giorno per la liberazione dei sindacalisti condannati in Birmania. Il destino della Birmania non riguarda solo la Birmania. Noi abbiamo ben presente il futuro geopolitico del mondo a partire dall'area asiatica ed il ruolo di grandi Paesi, come la Cina e l'India. Nella crescita economica di quell'area si colloca la Birmania, Paese ricco di risorse ma povero e stremato nelle sue energie. La prosperità della Birmania nell'economia e nella vita sociale è fondamentale per tutta l'Asia e solo il ripristino del diritto e della democrazia ed il rispetto dei diritti umani possono consentirle A noi sta a cuore il futuro della Birmania, come sta a cuore a tutti i Paesi e all'Organizzazione delle Nazioni Unite, e per questo motivo auspichiamo l'apertura di una nuova fase sul piano internazionale e sul piano interno. Sul piano internazionale, il nostro Paese ha concorso alla presentazione da parte dell'Unione europea di una risoluzione sulla situazione dei diritti umani in Myanmar, così si chiama la Birmania dal 1988, che è stata adottata dalla Terza Commissione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Recentemente, alla vigilia del quarto anniversario dell'arresto di Aung San Suu Kyi, l'Unione Europea ha adottato una dichiarazione con la quale si invoca il suo rilascio. Noi chiediamo che in tutte le sedi internazionali competenti, nel Consiglio di Sicurezza dell'ONU come nell'Unione europea, l'Italia si adoperi perché sia restituita la libertà ad Aung San Suu Kyi e si avvii una nuova fase interna, di dialogo tra le parti, le etnie e le organizzazioni sociali, per la transizione pacifica verso la democrazia attraverso un processo di riconciliazione. Sappiamo che in questo il ruolo di Aung San Suu Kyi è fondamentale. Nel 1995, a Pechino, alla quarta Conferenza mondiale delle donne promossa dall'ONU per l'uguaglianza, lo sviluppo e la pace, è stato affermato, nel nome di tutti i popoli, l'impegno delle donne perché sotto tutti i cieli i diritti delle donne fossero rispettati. Oggi facciamo nostro questo impegno per la liberazione di Aung San Suu Kyi. Una donna che esprime come poche la coscienza femminile democratica del mondo. In un'intervista di 11 anni fa a RAI Educational Aung San Suu Kyi ha manifestato tutta la sua straordinaria ricchezza umana e spirituale. Richiesta di indicare alcune opere particolarmente significative nella storia dell'umanità, Aung San Suu Kyi indicava i poemi indiani Ramayana e Mahabharata, la statua di Vishnu dormiente nella valle di Katmandu, la vetrata di Marc Chagall alle Nazioni Unite, la musica di Mozart insieme al canto gregoriano. Il valore di questa donna ci appartiene. Lei stessa spiega che a fondamento della sua azione c'è la fede buddista, con i suoi valori di verità, giustizia e compassione che, dice, "sono spesso i soli baluardi contro un potere inumano". Con queste premesse la politica di Aung San Suu Kyi non può che essere una buona politica. Una politica necessaria per la Birmania e per il mondo. Ed è per questo che pensiamo che ora vi possano essere le condizioni migliori per l'apertura di un dialogo vero in Birmania con il sostegno internazionale, che liberi il popolo e apra nuove prospettive di progresso e di unità. La via di Aung San Suu Kyi, di verità e di non violenza, è un patrimonio universale, inestimabile per l'intera umanità. Chiediamo oggi che il nostro Paese sostenga con nuove iniziative Aung San Suu Kyi e la Birmania democratica: chiediamo al Governo di attuare pienamente la risoluzione dell'ILO del 2000, di sostenere alla prossima riunione del Consiglio UE il rafforzamento della posizione comune dell'Unione Europea, inserendo anche le imprese del settore del legno nel blocco degli affari, di sostenere una risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU e di lavorare tenacemente perché la Cina e l'India, strategiche e fondamentali per questo obiettivo, modifichino la loro posizione. Chiediamo un impulso forte alle iniziative delle organizzazioni non governative e delle associazioni internazionali rivolte al popolo birmano. Per una libera iniziativa di parlamentari di entrambi gli schieramenti politici è sorta di recente nel Parlamento italiano l'associazione interparlamentare amici della Birmania che ha già avviato incontri, in particolare con Daw San San, responsabile della *National League for Democracy*, ed inviato una lettera al ministro degli affari esteri D'Alema. Signor Presidente, siamo certi che il dibattito di queste ore a seguito della mozione che abbiamo presentato segnerà un passo in avanti non solo per l'interesse generale della Birmania, ma per la coscienza democratica del mondo. Ovunque la libertà è offesa, limitata è la nostra libertà ad essere offesa e limitata. Ovunque cresce il dialogo democratico è la coscienza democratica del mondo che diventa più forte; ovunque si apre per un popolo la via della libertà, è la storia intera dell'umanità che è percorsa dal vento della libertà. E se è vero che ogni popolo ha la sua ora per la liberazione e il suo tempo di resistenza, oggi è più che mai vero che il tempo della libertà nel mondo globale è in ogni luogo, è per tutti, è per sempre. Il mio e il nostro auspicio è che il Governo italiano oggi esprima in ogni sede, con intelligenza e forza, questi sentimenti e questa volontà dell'Italia.

affari esteri*. L'Italia sta seguendo con grande attenzione ed apprensione gli sviluppi del quadro interno birmano, che ha subìto un preoccupante deterioramento dopo i disordini delle ultime settimane e gli arresti di numerosi esponenti dell'opposizione. Dopo le prime manifestazioni contro l'aumento del costo dei carburanti la Presidenza dell'Unione Europea ha diramato a nome nostro e di tutti i *partner* europei un comunicato di condanna, sollecitando il rilascio degli attivisti e l'avvio di un dialogo aperto ed inclusivo con tutte le componenti della società civile. La prima tappa della *road map* per la democrazia, varata dalla Giunta birmana nel 2003, la convenzione nazionale, si è conclusa il tre settembre, senza registrare alcun progresso sulla via del dialogo e della riconciliazione nazionale. I suoi lavori si sono chiusi senza indicazioni sui tempi dei prossimi passi: stesura della Costituzione, *referendum* costituzionale, elezioni. Il clima di tensione nel quale si sono svolti i lavori, la non inclusività del processo, l'assenza di un calendario sui seguiti ed i limiti evidenziati dal contenuto dei principi costituzionali sanciti dalla convenzione, concorrono a delineare un quadro delicato e controverso sul quale l'Italia manterrà, in stretto coordinamento con i *partner* dell'Unione Europea, un costante monitoraggio. Abbiamo effettuato proprio in questi giorni un passo presso l'ambasciata del Myanmar a Roma, al fine di esprimere la preoccupazione italiana per gli sviluppi della situazione del Paese e per ribadire la posizione comune raggiunta a Yangon dai rappresentanti UE. Una posizione con cui l'Italia ed i *partner* europei esprimono il proprio disappunto per il fallimento della convenzione nazionale, condannano il clima di repressione verificatosi in tutto il Paese nelle ultime settimane e richiamano il Governo di Myanmar al rilascio di tutti i prigionieri politici. Le attese della comunità internazionale sulla questione birmana sono in questa fase legate al mandato di buoni uffici del consigliere speciale del Segretario generale delle Nazioni Unite Ibrahim Gambari, che ha compiuto nei mesi scorsi un giro di consultazione nelle principali capitali interessate, in preparazione di una sua prossima missione a Yangon. L'Italia sostiene il mandato di Gambari, di cui condivide l'approccio costruttivo e «complessivo» che abbraccia tutti gli aspetti della problematica (inclusi i temi dell'aiuto umanitario, bambini e conflitti armati, lotta alla droga, obiettivi del Millennio, educazione, lavoro forzato, sanità). Anche in qualità di membri del Consiglio di Sicurezza intendiamo rinnovare il nostro supporto agli sforzi di Gambari favorendo il mantenimento di una posizione comune di pieno sostegno al suo mandato. La missione di Gambari si ispira agli stessi presupposti dell'iniziativa italiana «*Friends of the Bangkok Process*» (da noi rilevata dalla precedente *leadership* tailandese), improntata al dialogo critico e costruttivo con Rangoon, che nel novembre del 2005 ci ha visti promotori di un incontro a livello di alti funzionari al quale hanno partecipato rappresentanti europei, asiatici e - per la prima e sinora unica volta - un delegato del Myanmar. Riteniamo, infatti, che formule di dialogo critico costituiscano lo strumento più efficace per tentare di promuovere sviluppi in Myanmar. Una posizione di totale chiusura finirebbe invece per rafforzare l'auto-isolamento della Giunta ed arrecare ulteriori sofferenze alla popolazione civile. In questa ottica assume carattere prioritario la ricerca di un più stretto raccordo con i principali attori della scena birmana per compiere passi convergenti e trasmettere messaggi coerenti alla *leadership* di Yangon. Un ruolo chiave spetta ai partner asiatici, in particolare ai Paesi ASEAN, Cina e India, legate al Myanmar da interessi economici e strategici, che permettono a Pechino e a Nuova Delhi di esercitare un'influenza rilevante sulla Giunta. Anche l'ASEAN - su impulso in particolare di Filippine, Malesia, Indonesia e Singapore - ha gradualmente assunto toni meno concilianti verso il regime del Myanmar, esprimendo da ultimo forte preoccupazione per i più recenti avvenimenti. L'Italia si è costantemente adoperata in ambito UE e nelle altre sedi opportune per la liberazione di quella straordinaria donna che è Aung San Suu Kyi. Alla vigilia del rinnovo degli arresti domiciliari nel maggio scorso, l'Unione Europea ha adottato una dichiarazione ha adottato una dichiarazione per richiedere il rilascio della *leader* della Lega Nazionale per la democrazia e degli altri prigionieri politici. All'indomani della proroga, l'UE ha diramato un successivo comunicato esprimendo disappunto ed invitando il Governo birmano a rivedere la sua posizione in un'ottica di dialogo inclusivo, riconciliazione e cambiamento democratico. In materia di tutela dei diritti dell'uomo, l'Italia ha organizzato e finanziato, per il prossimo ottobre, la partecipazione di funzionari birmani ad un corso di formazione in diritto umanitario, diritti umani e diritto dei conflitti armati presso l'Istituto internazionale di diritto umanitario di Sanremo. L'adesione birmana alla nostra iniziativa costituisce per noi un significativo risultato anche alla luce della materia trattata, che interpretiamo come un segnale comunque positivo e come un riconoscimento per il nostro attivo impegno nella ricerca di un dialogo costruttivo con le autorità birmane. In ambito Nazioni Unite, lo scorso anno l'Italia ha attivamente concorso alla presentazione da parte della Unione Europea di una risoluzione su Myanmar, che è stata adottata dalla terza Commissione dell'Assemblea generale dell'ONU, nella quale abbiamo ottenuto l'inserimento di un esplicito richiamo al lavoro forzato. In gennaio abbiamo inoltre sostenuto la bozza di risoluzione proposta in Consiglio di Sicurezza dagli Stati Uniti, poi respinta a causa del veto posto da Cina e Russia. Nel dialogo con le agenzie internazionali registriamo il confortante esito delle missioni compiute nei mesi scorsi da alti funzionari ONU competenti in materia di bambini soldato e aiuto umanitario, nonché gli sviluppi relativi alla cooperazione con l'Organizzazione internazionale del lavoro, in particolare la firma, il 27 febbraio scorso, del protocollo d'intesa istitutivo di un meccanismo di denuncia che auspichiamo possa costituire un valido strumento nella lotta al lavoro forzato. L'Italia è molto sensibile ai bisogni della popolazione civile, è infatti opinione condivisa anche a livello UE che nel rispetto della posizione comune non si debbano risparmiare sforzi per lenire le sofferenze del popolo birmano e a tale scopo è unanime l'obiettivo di intensificare l'aiuto rivolto alla popolazione. Con questo spirito negli ultimi anni il Governo italiano ha promosso alcune qualificate iniziative volte a rispondere ai bisogni del popolo birmano, soprattutto in campo medico sanitario. Particolare attenzione è stata rivolta anche al problema della droga mediante interventi realizzati con l'UNODC. L'Italia intende continuare ad impegnarsi anche in qualità di membro del Consiglio di Sicurezza per la ricerca di soluzioni in grado di innescare una dinamica positiva nella questione birmana e di favorire un miglioramento della situazione sul piano dell'avvio di un autentico processo democratico aperto alla partecipazione di tutte le componenti della società birmana e della tutela dei diritti dell'uomo. Alla luce delle considerazioni che ho esposto, la posizione del Governo sulla parte dispositiva della mozione è la seguente. I paragrafi 1 e 3 sono accettabili. Come ho avuto modo di sottolineare, il Governo italiano è già fortemente impegnato nel tentativo di promuovere il rispetto dei diritti umani in Myanmar. Condivide quindi senza esitazioni l'incitazione a proseguire su questa strada. Proprio in questo spirito pienamente costruttivo, il Governo ritiene invece auspicabile un affinamento del paragrafo 2. In particolare: l'invito a promuovere un inasprimento della posizione comune della UE non è accettabile, in quanto tale inasprimento difficilmente produrrebbe dei risultati e rischierebbe invece di rafforzare l'autoisolamento della giunta, arrecando ulteriori sofferenze alla popolazione civile. L'Italia si è costantemente adoperata per ricercare un dialogo critico con le autorità birmane, sostenendo che formule di dialogo costruttivo, seppure fortemente critico, costituiscano lo strumento più efficace per promuovere sviluppi in Myanmar. Per questo riteniamo che gli obiettivi individuati dalla posizione comune rimangano validi e che si tratti piuttosto di adoperarsi per raggiungerli. Circa la parte relativa all'impegno del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e ad un'eventuale risoluzione, ho avuto modo di ricordare che questa strada è stata già percorsa, senza successo, nel gennaio scorso. Purtroppo, in quell'occasione, una risoluzione, anche da noi sostenuta, ha incontrato il veto di Cina e Russia. In questa fase, è preferibile tentare altre vie, per evitare di scontrarsi con gli stessi problemi. Più proficuo potrebbe rivelarsi, in particolare, assicurare un pieno sostegno ad un'azione più efficace del Segretario Generale delle Nazioni Unite. Pertanto, il paragrafo 2 è accettabile nella seguente riformulazione: «ad adoperarsi per il raggiungimento degli obiettivi indicati dalla posizione comune della UE e a sostenere l'impegno e gli sforzi del Segretario generale delle Nazioni Unite nei confronti della situazione in Myanmar, sostenendo ugualmente le iniziative in tal senso nelle istanze delle Nazioni Unite e, qualora ne esistano le condizioni, anche in Consiglio di Sicurezza».

Signor Presidente, intervengo, a nome del Gruppo Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti Italiani, per esprimere il nostro voto favorevole, anche se ci saremmo aspettati pieno accoglimento da parte del Governo di questo atto di sindacato ispettivo. Colgo anche l'occasione per aggiungere la mia firma a questo atto di sindacato ispettivo, che probabilmente mi era sfuggito,

che ha imposto l'arbitrio come legge e come modalità di governo. Va anche ricordato che esiste una campagna in favore della Birmania lanciata nel nostro Paese da un sindacato, la CISL, ma anche da associazioni e organizzazioni

sui *media* e all'attenzione dell'ordine pubblico proprio per la violenta censura interna che viene esercitata da quello che di fatto è un regime.

Del Nobel per la pace abbiamo già parlato, ma bisogna parlare anche delle centinaia di migliaia di uomini, donne e bambini tuttora costretti al lavoro forzato da parte sia dei militari che delle autorità locali, persone spesso obbligate a deportazioni forzate in un Paese in cui sono comuni la detenzione, le esecuzioni, le torture, gli stupri che vengono utilizzati come mezzi di potere. Nonostante questo, le associazioni della vita civile, compresi i sindacati (va ricordato che il sindacato birmano, l'FTUB,

militare. Da questo punto di vista, accanto alle violazioni dei fondamentali diritti umani e del lavoro - anche a questo ha dato risalto la senatrice Soliani - vi è pure la gravissima violazione dei diritti ambientali: la distruzione e il taglio illegale delle foreste di tek, il dissennato sfruttamento minerario, la costruzione delle dighe sul fiume Salween che ridurranno alla povertà oltre 500.000 contadini e pescatori,

perché la storia, la politica ci insegnano che tutti i boicottaggi di tipo economico e culturali adottati nei confronti di altri Paesi hanno sempre comportato il peggioramento della vita e delle condizioni delle persone che vivono in quei Paesi, soprattutto dei bambini.

ad esempio, nei confronti dell'Iraq, oppure nei confronti di Cuba e di altri Paesi. Chiediamo però che questa posizione venga tenuta anche nei confronti di tutti gli altri Paesi

quindi, che da parte del Governo vi debba essere una presa di posizione chiara all'interno di tutti gli Organismi internazionali, come viene chiesto dall'atto ispettivo presentato dalla senatrice Soliani, senza timori,

signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, parliamo oggi di un Paese straordinario, tra i più belli e affascinanti al mondo, eppure un Paese nel quale il popolo drammaticamente vive da oltre 50 anni sotto una dittatura militare durissima in cui sono negate le più elementari libertà politiche e sindacali: come è stato ricordato, Aung San Suu Kyi dal 2003 è nuovamente agli arresti, 92 deputati di quel Paese sono da anni in esilio e solo ultimamente sei sindacalisti, semplicemente per avere organizzato il 1° maggio scorso un seminario sui diritti sindacali, sono stati condannati a 28 e 20 anni di carcere, in cui un sindacalista, Myo Aung Thant, da 10 anni è in prigione ed è stato condannato all'ergastolo solo perché sindacalista. Un regime militare basato sul lavoro forzato, sull'uso massiccio del lavoro forzato, sulle deportazioni di massa, sull'uso di bambini soldato, sul traffico di oppio e metanfetamine, sull'esercizio della violenza sistematica nei confronti delle donne. Ma la discussione che svolgiamo oggi è però attualissima, visto che proprio nei giorni scorsi quel regime è stato scosso ed ha reagito con una durissima repressione nei confronti di lavoratori e cittadini

avvenuti intorno al 15 agosto e che hanno portato nei giorni scorsi al fermo di oltre 150 persone. L'opinione pubblica italiana da tempo segue con attenzione le sorti di quel Paese, le sofferenze di quel popolo. Proprio ieri i sindacati CGIL, CISL e UIL hanno approvato un ordine del giorno per la libertà dei sindacalisti arrestati e condannati e per l'avvio di un processo che porti alla libertà sindacale e di manifestazione. Io credo, a nome del Gruppo Sinistra Democratica per il unanime di questa mozione oggi nell'Aula del Senato possa impegnare ancor di più il Governo, che si è espresso nelle parole del sottosegretario Di Santo, a moltiplicare gli sforzi in tutte le sedi internazionali, a partire dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Ho ascoltato le considerazioni del Sottosegretario, ma anche su altre materie ci siamo trovati a doversi scontrare con difficoltà, veti, obiezioni da parte di altri componenti del Consiglio di Sicurezza: ricordo tra tutte la moratoria delle esecuzioni capitali. Ma questo non ci esime dal continuare e dal tentare ancora, dall'insistere in tutte le sedi internazionali perché si arrivi alla liberazione di Aung San Suu Kyi; perché si affermi il rispetto dei più elementari diritti umani, di quelli politici e sindacali; perché si attui pienamente la risoluzione dell'ILO (l'Organizzazione internazionale del lavoro) del 2000, contro il lavoro forzato; perché si rafforzino tutti i controlli e le iniziative affinché non si aggiri l'embargo per le forniture di armi del regime di Rangoon, previsto dalla posizione comune dell'Unione Europea. Vorrei ricordare al Sottosegretario che, secondo un rapporto di Amnesty International, il Governo indiano sta trasferendo alla giunta militare birmana degli elicotteri d'attacco, che hanno anche delle componenti prodotte in Italia. Dobbiamo rafforzare, da questo punto di vista, l'azione perché non si aggiri in nessun modo l'embargo per la fornitura di armi, appunto previsto dalla posizione comune dell'Unione Europea; affinché anche il popolo birmano, con il contributo della comunità internazionale, possa vivere senza più gli orrori che ha conosciuto e subìto nel corso degli ultimi cinquant'anni.

l'ardore ed il coraggio di presentare e che abbiamo anche voluto aggiornare, visti appunto i recenti ed ultimi sviluppi. E lo faccio con grande convinzione, con la convinzione mia e delle colleghe e dei colleghi, che già dalla scorsa legislatura hanno lavorato alacremente per seguire la situazione birmana, incontrando rappresentanti dei movimenti sindacali del Governo birmano in esilio e presentando, maggioranza ed opposizione, ben due risoluzioni e mozioni, che sono state discusse e mai inspiegabilmente votate dall'Aula. Quindi, oggi, colmiamo anche un ritardo e faremo in modo che le dichiarazioni ed il pronunciamento del Senato si vadano ad aggiungere a quello di altri organismi parlamentari, alle richieste ed alle sollecitazioni che ci provengono dal Governo birmano in esilio, dai movimenti sindacali. In particolare, vorrei ricordare il ruolo importante della CISL in questa campagna e di tutti coloro che hanno a cuore la libertà ed i diritti umani in quel Paese. Ho conosciuto personalmente il dramma birmano ben dieci anni fa, incontrando a Chiang Mai in Thailandia i rappresentanti dell'esercito di liberazione Karen. Erano giovani studenti universitari che mi raccontarono il dramma che vissero nel 1988, quando la giunta militare non esitò a sterminare quegli studenti che stavano manifestando pacificamente.

un Paese che vive, ormai da decenni, una tragedia, senza che la comunità internazionale riesca a scalfire significativamente la protervia e la crudele determinazione del regime militare che tiene appunto quel popolo sotto un pugno di ferro. È un regime, questo, che oggi purtroppo, va constatato, riesce a giovarsi di un complicato intreccio di relazioni politiche ed economiche e di un rinnovato interesse geostrategico alle sue risorse naturali. La Cina e l'India oggi si contendono una posizione privilegiata verso la Birmania, la Cina stringendo accordi multimiliardari per lo sfruttamento del gas naturale e l'India facendo altrettanto, però cercando di agevolare l'esportazione, soprattutto di armi. Addirittura la Corea del Nord ha riaperto le relazioni diplomatiche dopo anni e anni di gelo.

una cattedrale nel deserto, che la dice lunga anche su come la giunta militare voglia continuare a mantenere saldo nelle sue mani il potere. Come ha detto il senatore Iovene, anche noi abbiamo delle responsabilità perché, proprio grazie alle maglie larghe delle normative europee sull'esportazione di armamenti in Paesi terzi, oggi ci troviamo di fronte a una situazione paradossale nella quale un elicottero prodotto in India con componenti europee, tra cui italiane, verrà esportato in Birmania e verrà utilizzato da quell'esercito e da quel Governo per continuare nella sua opera di repressione, in un Paese dove il 40 per cento del bilancio dello Stato viene assorbito dalle spese militari e, per contro, solo lo 0,3 per cento viene speso per l'assistenza sanitaria, mentre quello stesso Paese vede migliaia e migliaia di persone cadere malate di AIDS, di malaria o di tubercolosi. poi un accordo che l'Italia ha concluso con l'India per la cooperazione nel settore della difesa. Noi ci siamo astenuti su quell'accordo, proprio perché vedevamo un rischio enorme, poi confortato dalle denunce di Human Rights Watch, di un allentamento del controllo della legge n. 185 del 1990, della possibilità che anche sistemi d'arma italiani o coprodotti possano andare a finire in Birmania; purtroppo il caso, la storia e l'evidenza ci hanno dato ragione. Stretto quindi da giochi d'interesse geopolitico e geostrategico e dalla retorica dell'esportazione della democrazia, che non ci appartiene, il popolo birmano continua a soffrire. Soffre della repressione spietata scatenata dopo le recenti proteste causate dall'aumento indiscriminato dei prezzi del carburante, che ha portato all'aumento notevole dei prezzi del cibo e dei trasporti pubblici. Oltre 2,5 milioni di birmani ogni giorno si muovono con i trasporti pubblici e oggi devono spendere il 90 per cento del loro salario soltanto per comprarsi il cibo.

Il reddito *pro capite* è di 225 dollari l'anno e ben il 90 per cento della popolazione vive sotto la soglia della povertà. Questo è un paradosso, perché la Birmania, come è stato anche detto prima, era considerato uno dei Paesi più ricchi dell'Asia, soprattutto per la produzione agricola ma anche ora per l'enorme disponibilità di risorse naturali, tek, pietre preziose, gas naturale. Invece i fondi che arrivano alla giunta militare birmana anche dallo sviluppo dell'industria turistica (ci tengo molto a dirlo perché è un'industria che oggi è piagata dal lavoro schiavo)

Un Paese che soffre la fame, la repressione, il lavoro schiavo e la violenza sessuale, lo stupro usato come arma di dissuasione militare e politica. Soffre nella persona del suo *leader* spirituale, appunto Aung San Suu Kyi, premio Nobel per la pace, che ha passato undici degli ultimi diciassette anni agli arresti domiciliari, e che soffre nel vedere i *leader* dei movimenti che hanno coordinato le ultime proteste, il cosiddetto Movimento 88, arrestati, alcuni torturati (uno morto sotto le torture), constatare anche che, nonostante le pressioni internazionali, la giunta sta preparando il campo alla sua permanenza al potere. In questa discussione è mancato al fatto che, contemporaneamente alle proteste per l'aumento del carburante, la giunta militare ha chiuso un processo illegittimo, non trasparente, non democratico, che porterà, se non vi sarà una responsabilità seria da parte della comunità internazionale per disconoscere tale processo, ad adottare una Costituzione che rafforzerà il potere dei militari, escluderà i partiti democratici e quindi perpetuerà il potere purtroppo, rappresenta un notevole passo indietro rispetto a quanto il Parlamento europeo, proprio qualche giorno fa, ha esplicitamente raccomandato in termini di rafforzamento della posizione europea, chiedendo anche all'Italia di adoperarsi, insieme agli altri Stati membri del Consiglio di Sicurezza, per una nuova risoluzione vincolante. Non vorremmo che in questo caso le ragioni della diplomazia prendessero il sopravvento rispetto a quelle della politica, di un impegno che questo Governo ha preso nei confronti della Birmania e che, a nostro parere, dev'essere ulteriormente rafforzato e confermato.

Vorrei sottolineare, nell'esprimere questo nostro voto, due punti principali. In primo luogo, ringrazio i colleghi che hanno particolarmente sostenuto questa mozione per aver portato all'attenzione, focalizzandolo su un Paese,

È importante sottolineare questo aspetto. Oggi ci occupiamo della Birmania: sappiamo bene, credo, che i diritti umani sono conculcati in molti altri Paesi e che, dopo un periodo in cui c'è stata una tendenza positiva

così costantemente e direi acriticamente vicino alla giunta militare birmana, che ha perpetrato tutto quanto abbiamo sentito nel corso di questa discussione. La Repubblica popolare cinese è di gran lunga il primo *partner* commerciale della Birmania: è un importante *partner* commerciale anche per Paesi assai più lontani, come per esempio il nostro, figuriamoci per la Birmania, e di conseguenza, fosse anche solo per questo, ha già forti responsabilità. Ma non si tratta solo di una responsabilità di relazioni commerciali: vi è un sostegno politico che, come dicevo, ha ben

Unite una risoluzione a favore dei diritti umani della Birmania ha incontrato (guarda caso) il veto di Russia e Cina. Sappiamo dunque chi è che potrebbe davvero esercitare reali pressioni sulla Birmania. È stato sostenuto che i boicottaggi economici hanno generalmente scarso successo e spesso peggiorano la situazione di

ci suggerisce che, se il primo *partner* commerciale della Birmania non soltanto non partecipa al boicottaggio, ma sostiene attivamente, specialmente dal punto di vista militare, questa giunta, difficilmente un'azione di carattere economico da parte di altri Paesi potrà

Ritengo quindi che sia importante non dimenticare che cosa c'è dietro e accanto alla giunta militare birmana; essa non è una monade indipendente che non ha sostegno all'estero. Ciò bisognerebbe ricordarlo tenendo presente che fra undici mesi si celebreranno le Olimpiadi a Pechino, che saranno una colossale operazione di propaganda a favore di un regime dittatoriale, che a suo sua volta sostiene altri regimi dittatoriali.

il dispositivo di questa mozione. Credo che non dovremmo restare indietro rispetto ad altri, in particolare rispetto all'Unione Europea, nel sostenere azioni forti o quantomeno azioni simboliche presso le Nazioni Unite nei confronti della giunta militare, della feroce dittatura che c'è in Birmania. Pertanto, il voto sarà favorevole, con il rammarico che la mozione è stata